di senatore, e anche di europarlamentare. La figura di Maurizio Valenzi può essere ricordata per tante ragioni. La prima che da cittadina napoletana voglio ricordare è stata la sua lunghissima esperienza come sindaco di Napoli. Per otto anni ha guidato la difficile e bellissima città di Napoli, otto anni in cui ha dovuto affrontare anche problemi gravissimi: innanzi tutto lo scoppio dell'epidemia di colera

e tenendo a dire che il suo era un bilancio più che attivo, tanto da apporre alla storia della propria vita, pubblicata poi dall'editore Pironti, il titolo «Confesso che mi sono divertito». Maurizio Valenzi è una figura anche storica del comunismo e della Resistenza del nostro Paese: ha fatto parte del gruppo dei comunisti napoletani

Maurizio Valenzi non è stato solo un uomo politico legato per molti anni e anche molto amichevolmente al Presidente della Repubblica, che pochi giorni fa

È sempre appartenuto al Partito Comunista Italiano, fin dal ritorno in Italia di Palmiro Togliatti. Grazie, il tratto di amore per la propria città e di umanità, con il quale egli ha avuto modo di affrontare anche responsabilità difficili. In qualche modo Valenzi è stato un sindaco di Napoli fin troppo unanimistico nella ricerca di collaborazioni; molti dei problemi di Napoli non è riuscito a risolverli, ma la sua generosità e la sua simpatia umana fanno sì che in un'assemblea politica non si possa che ricordarlo se non con straordinario affetto e simpatia

banale, anche se certamente di difficile applicazione, perché una copertura sui cosiddetti tre saldi sarebbe assolutamente più rigorosa, soprattutto nei momenti di difficoltà.

tenta di sottolinearne nuovamente al Governo e al relatore il rilievo. Esso è volto ad introdurre nella legge di contabilità un principio - non si tratta di niente di più a mio giudizio estremamente rilevante. Capita spesso che, quando valutiamo la sussistenza della copertura finanziaria di una nuova disposizione di legge che produce degli oneri (e per questa ragione ha bisogno di copertura),

Capita molto spesso però che da una norma che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato derivino oneri di carattere finanziario molto significativi

quando lo Stato - me lo faccia dire in modo semplice - complica la vita alle imprese attraverso una nuova legge che impone adempimenti burocratici onerosi in capo alle imprese, una valutazione di questi oneri aggiuntivi per gli operatori economici deve essere contenuta nella relazione tecnica che

sotto il profilo delle politiche fiscali, si tenga conto di questo onere aggiuntivo che l'innovazione legislativa pone in capo alle imprese. Quante volte in questa sede, colleghi, ci siamo soffermati sul fatto che gli appesantimenti burocratici si moltiplicano? Recentemente c'è stato uno studio commissionato a un importante istituto di ricerca da una grande organizzazione degli artigiani, la Confartigianato, che dimostra che gli appesantimenti burocratici, con relativi oneri per le imprese, hanno un rilievo economico enorme per lo sviluppo economico del Paese nel suo complesso. Noi vorremmo limitarci ad introdurre nella legge di contabilità un principio ispiratore: quando lo Stato, rendendo onerosi certi adempimenti, complica la vita alle imprese, imprese, deve riconoscere l'esistenza di quell'appesantimento e in qualche misura farne cenno all'interno della relazione tecnica, in maniera tale che la politica fiscale

mi pronuncerei nello stesso senso del relatore, vale a dire che un ordine del giorno sarebbe accoglibile. Il testo, così com'è, è assolutamente interessante e colpisce la sensibilità di molti di noi;

è stato un ampio dibattito, che si è dipanato in anni e anni di lavori parlamentari, sulla considerazione degli effetti indiretti sullo sviluppo dell'economia delle misure di carattere fiscale, la cosiddetta curva di Laffer applicata alla finanza pubblica. È una una valutazione assolutamente interessante da un punto di vista teorico e anche pratico, ma fino ad ora non si è mai acceduto a questo tipo di impostazione, perché il calcolo degli effetti indiretti è a volte una prova quasi diabolica, essendo difficilissimo da fare.

com'è noto, nella redazione dei provvedimenti di carattere governativo è indispensabile avere una relazione sugli effetti amministrativi e quindi anche, indirettamente, sugli oneri. Sotto questo profilo, la proposta si potrebbe condividere e penso che del giorno sia uno strumento migliore, piuttosto che una definizione normativa che sarebbe, credo, troppo vincolante e rischierebbe di creare difficoltà pratiche molto serie all'attività legislativa. Pertanto, nel condividere assolutamente lo spirito, faccio presente che però questo può avere effetti controproducenti, perché ogni principio va applicato estensivamente e non si può applicare solo ad una fattispecie; quindi se riconosciamo gli effetti indiretti, dobbiamo riconoscerli in tutte le fattispecie e questo avrebbe qualche difficoltà applicativa. Tuttavia, sotto un profilo conoscitivo, sicuramente non vi è difficoltà a riconoscere la bontà dell'approccio lumeggiato nell'emendamento in questione.

non posso accogliere l'invito a trasformare questo emendamento in ordine del giorno. Faccio notare al vice ministro Vegas che il testo dell'emendamento parla esplicitamente di un contenuto della relazione e non del testo di legge

Detto questo, penso sia necessario votare perché invece, secondo me, sarebbe assolutamente positivo introdurre questo principio generale in norma e invito i colleghi, che

Presidente, dichiaro il voto contrario del Partito Democratico su questo emendamento per una ragione che,

del riferimento a possibilità di rimodulazioni tra programmi, ma all'interno della stessa missione, non c'è dubbio che il difetto fondamentale - quello che era, a mio giudizio, una ragione di contrarietà molto robusta alla alla proposta del Governo - viene meno. Tuttavia vorrei invitare il Governo e il relatore a valutare valutare che c'è un'altra differenza tra i due testi che, attraverso la proposta di integrazione avanzata dal relatore sul testo del Governo, non viene risolta;

cerchiamo di andare all'essenziale, malgrado il carattere esoterico del testo che abbiamo di fronte - che riguarda sostanzialmente la flessibilità nella gestione riconosciuta al Governo all'interno dei programmi e, in ogni caso, tra programmi della stessa missione. Nel testo del Governo il riferimento ad un'identica missione non c'era, mentre adesso, con la proposta del relatore che il Governo ha accettato,

sono variazioni compensative, anche se mi sembra ovvio che non possono peggiorare i saldi, perché ciò è impedito da un'altra parte della legge di contabilità che stiamo votando. Si potrebbe però trattare di interventi del Governo nel corso d'anno che non abbiano carattere compensativo. In quel caso, la decisione di bilancio assunta dal Parlamento verrebbe modificata in modo, secondo me, inaccettabile. Se Se il testo del Governo viene riformulato in modo da introdurre il principio della compensazione tra le variazioni,

Grazie, nel testo con l'approvazione di emendamenti - in questo caso in Commissione, non in Aula - una delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa sulla base di alcuni principi e criteri direttivi. L'emendamento 42.100, che non considero essenziale ma che a mio giudizio sarebbe utile, si limita ad aggiungere qualche principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega nella fase che si aprirà immediatamente dopo l'approvazione da parte del Parlamento del Parlamento di questo disegno di legge. In particolare, tale proposta tende a definire con maggiore puntualità i margini di i margini di operatività riconosciuti nel campo della gestione ad ogni dirigente della pubblica amministrazione responsabile di programma, sia dal punto di vista della necessità che renda conto, sia dal punto di vista della necessità che mi si passi l'espressione - tenga conto, e cioè monitori in maniera molto puntuale, di giorno in giorno, di fase in fase, l'attuazione del bilancio per quello che riguarda lo specifico programma di spesa affidato alla sua responsabilità. Si tratta, quindi, di un emendamento che naturalmente si può

aderirei alla proposta, perché nell'emendamento è contenuta semplicemente una specificazione di cui si può tener conto nella fase dell'esercizio della delega e, in questo caso, sia che si tratti di un ordine del giorno o di una norma di legge non cambia moltissimo, giacché sono certo che lo spirito con cui il Governo eserciterà la delega sarà perfettamente coerente con questo emendamento. PRESIDENTE. Il restante

stando al calendario vigente, il Documento di programmazione economico-finanziaria attuale verrà comunque presentato secondo la vecchia legge,

52.150 serve proprio a definire i termini della nuova materia e quindi a regolamentare i nuovi atti che verranno in applicazione della legge che stiamo votando.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, non molto tempo fa (nel mese di giugno dello scorso anno) nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica degli anni 2009-2013, veniva annunciata la strategia del Governo con queste testuali parole: «Interrompiamo la tradizione di discussioni che sulle finanziarie, per prepararle, per farle e per controllarne infine gli effetti occupavano ogni anno mediamente nove mesi su dieci. All'opposto, il nostro piano sarà anticipato entro l'estate e stabilizzato, proiettandolo sull'arco di un triennio, per creare solide basi per la vita economica». Sappiamo tutti come è andata a finire: la manovra finanziaria messa in campo l'estate scorsa e presentata come un'innovazione nella sessione di bilancio, in termini di anticipazione e programmazione triennale, ha dimostrato oggi tutti i suoi limiti.

Perché, come dicevo, delle due cose l'una: o il Governo a giugno non aveva intuito la gravità della crisi economica e non si era preparato ad adottare misure efficaci - il che, di per sé, sarebbe grave - oppure l'utilizzo contraddittorio di risorse pubbliche che ha segnato le scelte di questo Governo appare ancora più ancora più irresponsabile. Siamo quindi passati dalle leggi finanziarie omnicomprensive del passato a una manovra economica inconcludente, che continua e si trascina da oltre nove mesi. È un fatto certamente grave, non solo per la trasparenza e l'approfondimento del processo di formazione del bilancio dello Stato, ma anche perché - ed è un fatto ancora più grave, anzi gravissimo - in un momento di crisi drammatica il Governo rinuncia ad avere oggi una linea di politica economica credibile, capace di affrontare una disparità vergognosa che si sta sempre più determinando nelle condizioni sociali della nostra gente e del nostro Paese. Ricordo questo aspetto non trascurabile della storia recente per riportare un po' di realismo su un'eccessiva enfasi che sta riguardando alcuni principi richiamati in questo disegno di legge, come semplificazione, armonizzazione, razionalizzazione e flessibilità. In realtà, resta per noi un problema politico di fondo: nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, nella definizione, che non è solo tecnica, dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche, resta difficile un'efficace valutazione della portata delle novità in esso contenute, così come ogni possibilità di prevedere un successo reale che le stesse potranno ottenere nella loro attuazione, se prima non viene definito e attuato un sano equilibrio tra la piena responsabilità del Governo nel definire le scelte economiche necessarie al Paese e il potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio. si evidenzia una prima nostra forte preoccupazione perché nel dibattito, sempre attuale, relativo ad una moderna riforma della Costituzione sta pericolosamente penetrando, invadendo e condizionando l'intera legislatura il progetto politico di creare le condizioni giuridiche per un Governo forte. L'idea di un Esecutivo decisionista corrisponde infatti alla pratica quotidiana di questa legislatura, che in dieci mesi ha visto oltre 70 volte il ricorso a decreti, rispetto ai quali il Parlamento ha avuto una funzione di mera registrazione contabile e notarile. Dobbiamo fare attenzione! Se prima la crisi economica ha accentuato in molti Paesi la tendenza a rafforzare gli Esecutivi, ad attenuare il ruolo dei Parlamenti e a percorrere procedure legislative rapide per rispondere alle notevoli emergenze, le prime verifiche sulla qualità delle risposte politiche alla crisi stessa hanno messo in luce i molti limiti dei Governi forti, perché rapidità di esecuzione ha significato molto spesso rapidità di errore. La prospettiva disegnata in questo progetto di legge è certamente coerente con l'evoluzione più recente della finanza pubblica italiana in virtù, da un lato, degli impegni contratti dal nostro Paese in sede europea, codificati nel Patto di stabilità e crescita dall'altro, della riforma in senso federale dell'ordinamento dello Stato, in particolare con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle autonomie territoriali. Questo progetto di legge trova una sua altrettanto coerente ragione in due punti di debolezza del passato che ci trasciniamo da troppi anni: economico-finanziaria, che avrebbe dovuto definire gli orientamenti macroeconomici ed individuare gli obiettivi relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione, stabilendo il relativo fabbisogno del settore statale, rimaneva lettera morta dopo lunghissime discussioni parlamentari perché,

i cosiddetti tagli di spesa su cui si concentra la discussione delle varie leggi finanziarie non possono che influire sul 5 per cento delle uscite già previste in bilancio. E qui, signora Presidente, emerge la seconda nostra forte preoccupazione. Abbiamo apprezzato lo sforzo di razionalizzazione espresso dal provvedimento in esame. Abbiamo apprezzato il lavoro guidato dal presidente Azzollini in Commissione bilancio. Ma in considerazione del fatto che sono diverse le problematiche per le quali sono previste deleghe legislative - mi riferisco agli articoli 2, 30, 49 e 50 - restano aperte molte questioni, alcune per noi irrisolte. La prima: l'indicazione della pressione fiscale complessiva. Non ci convincono le motivazioni addotte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, secondo cui deve essere il cittadino elettore a giudicare come il Governo e la sua maggioranza avranno proposto la coppia beneficio-sacrificio. Noi riteniamo necessario invece definire nella Decisione quadro di finanza pubblica il limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale dei tributi e contributi ed il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici, assicurando il rispetto di tale limite e definendo di conseguenza, con il coinvolgimento della Conferenza unificata, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Diciamo questo in coerenza col dispositivo dell'ordine del giorno approvato dal Senato in sede di esame della legge sul federalismo fiscale, laddove si è rilevato che la pressione fiscale complessiva, riferita all'anno 2006, è stata del 40,6 e nel 2008 tale quota è salita fino al 43,3 per cento e che l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento del rapporto deficit-PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti rivolgo a lei, presidente Azzollini: riteniamo necessaria la presentazione di una relazione sui risultati della lotta all'evasione fiscale, come allegato alla relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, per consentire al Parlamento la disponibilità di informazioni costantemente aggiornate. Non a caso, nella Nota informativa 2009-2011 sugli andamenti di finanza pubblica, presentata dal Governo nel febbraio scorso e che non ha ricevuto un'adeguata attenzione, vi è una stridente incongruenza tra le previsioni del quadro macroeconomico e le previsioni sulle entrate. In particolare mi riferisco al gettito per le imposte indirette, al quale l'analisi dei dati ufficiali porta a concludere che la perdita prevista dal Ministero dell'economia va molto oltre gli effetti dovuti alla recessione in corso. E si registra un ampliamento dell'evasione fiscale di 13 miliardi nel 2008, 16 miliardi nel 2009, 14 miliardi nel 2010. La terza questione è che questa legge di riforma rischia di diventare un'opera incompiuta, e lo spiega con grande competenza e professionalità il sottosegretario Vegas in un pregevole e recente libro dal titolo "Il bilancio dello Stato", laddove, sulle prospettive di riforma, scrive testualmente che "la modifica della struttura dei documenti di bilancio e della legge finanziaria dovrebbe essere seguita da una più ampia modifica dei Regolamenti parlamentari, alla stregua della considerazione che le attuali procedure non hanno sortito gli effetti virtuosi, come dimostra il fatto che il deficit ed il disavanzo sono cresciuti malgrado l'esistenza di norme regolamentari che tendevano ad impedirlo". sulla scelta che adotteremo in merito alla nuova configurazione della manovra finanziaria, occorrerà comunque consolidare, migliorare e rafforzare il ruolo da assegnare al Parlamento, non solo nella fase di approvazione del bilancio, ma anche in quelle a questa successiva, e questo sia nella direzione di un esame più approfondito del disegno di legge di rendiconto sia nella direzione di attivare procedure efficaci e trasparenti azioni di monitoraggio costante dell'andamento della spesa pubblica. Per questo, in attesa di quanto verrà fatto in seconda lettura alla Camera dei deputati, il voto dell'Italia dei Valori sarà un voto realistico e comprensibile di astensione.

sia ai cambiamenti istituzionali, quali l'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria e la riforma federale della Repubblica, che alle condizioni dei conti pubblici. La necessità di contenere il disavanzo senza ulteriori aumenti della pressione fiscale richiede infatti un'attenta pianificazione ed un controllo della spesa, così come l'esiguità delle risorse ne impone un utilizzo efficiente, ponendo attenzione particolare ai risultati dell'azione pubblica mediante un adeguato sistema di indicatori che consenta di monitorare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche. La riforma in esame è frutto di un'ampia convergenza tra maggioranza ed opposizioni. Ciò non è dovuto al fatto che si tratta di una legge meramente tecnica ad esclusivo appannaggio di pochi addetti ai lavori, come si potrebbe erroneamente pensare. Al contrario, essa ha una grande e forte valenza politica: trova infatti nella Costituzione, segnatamente all'articolo 81, e più in generale nel nevralgico rapporto tra Governo, Parlamento e cittadini, il suo principale fondamento. Si intende con essa riallocare il potere decisionale e di controllo sul bilancio a favore di una rinnovata dialettica tra Governo, Parlamento e cittadini. Ad oggi infatti gran parte dell'attenzione si rivolge e si esaurisce sulla legge finanziaria, ovvero sullo strumento che serve tendenzialmente alla riduzione del deficit. Ciò appare un'evidente stortura, in quanto, al contrario, è il bilancio che rappresenta la parte rilevante delle spese. Concentrarsi quindi su di esso appare una regola di buon senso. Se lo si vorrà, la riforma in esame permetterà agli attori istituzionali di indirizzare l'attenzione sulle grandi componenti del bilancio, evidenziandone, e qui ne emerge la portata politica, scelte e responsabilità di natura politica. Conseguentemente, un miglioramento della legge di bilancio determinerà anche un miglioramento delle scelte di prelievo e di quelle allocative, anche attraverso l'aumento della trasparenza e dei sistemi di controllo. Infatti, se con il provvedimento all'esame dell'Aula si è voluto riconoscere un maggiore livello di flessibilità al Governo, dall'altro canto si è ritenuto opportuno aumentare la quantità e la qualità del controllo. il provvedimento in esame testimonia un importante cambiamento culturale, nato dalla scarsa soddisfazione maturata - non solo nel nostro Paese - nei confronti dei controlli di legalità, che ha portato a sostituire, nella gestione delle risorse pubbliche, il controllo sulle procedure con un approccio basato sui risultati. Il Parlamento rinuncia ad un controllo di legalità sui singoli atti di gestione del Governo a favore della valutazione dei risultati e dell'impiego delle risorse pubbliche mediante l'introduzione di un sistema di indicatori di *performance* confrontabili, basato su principi e metodologie comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, e la realizzazione di un programma di analisi e valutazione della spesa. Il bilancio diventa quindi lo strumento più diretto per misurare i risultati. Ciò concorre a migliorare la definizione degli obiettivi e i controlli sui risultati, a migliorare la programmazione e la qualità del *management*, la trasparenza e l'allocazione delle risorse, nonché a promuovere una disciplina fiscale più efficiente. Altrettante sono tuttavia le criticità legate ad una cultura fortemente orientata al risultato, alla selezione degli indicatori di *performance*, alla carenza dei dati; spesso gli indicatori scelti descrivono l'attività che le pubbliche amministrazioni svolgono e non i risultati che ottengono. Il successo dipende dall'individuazione di sistemi incentivanti. Inoltre, gran parte della spesa pubblica avviene a livello di governo locale richiedendo un coinvolgimento dei sottolivelli di governo rispetto ai quali la capacità del Governo centrale di monitorare le *performance* e di incidere sui meccanismi di miglioramento è minore. A fronte della rinuncia del Parlamento al controllo di legalità e alla riconosciuta maggiore flessibilità del Governo, era necessario quindi determinare una responsabilizzazione, un contrappeso. Condividiamo particolarmente quindi le modifiche introdotte in Commissione ed in Aula, grazie al contributo delle opposizioni, volte a riconoscere maggiori strumenti di controllo al Parlamento, criteri condivisi di nomina del Presidente dell'ISTAT, criteri migliori per la definizione del Patto di stabilità interno e, da ultimo, per quanto ci riguarda, garanzie che le procedure di controllo della spesa pubblica e di controllo del Patto di stabilità, quindi anche dei livelli di rispetto della finanza europea, avvengano, per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, nel rispetto delle prerogative autonomistiche e delle procedure previste dagli Statuti speciali. si articolano nel Titolo II, dedicato nella sua interezza alla trasparenza e al controllo della spesa e si sostanziano in particolare nell'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, nella Struttura unica di supporto tecnico che dovrà fornire gli elementi funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica e nell'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile. Al Parlamento sarà garantita quindi massima accessibilità all'informazione. Tutto ciò creerà un rinnovato rapporto dialettico tra Governo e Parlamento e anche con i cittadini. È ovvio che, come dicevamo prima, il limite che scontiamo anche in questa riforma è dato dalla circostanza che il controllo parlamentare è però attenuato sia con riferimento alla nuova riforma riforma introdotta, che riguarda il federalismo fiscale, sia per quanto riguarda il controllo dei conti pubblici degli enti locali. Siamo tuttavia soddisfatti del risultato raggiunto, ove si consideri tutto ciò creerà un rinnovato rapporto virtuoso tra Governo e Parlamento e una maggiore trasparenza nelle scelte di bilancio, nel rapporto e nella accessibilità a queste scelte da parte dei singoli cittadini. Infatti, in ossequio ai principi di analisi e valutazione della spesa, lo Stato sarà chiamato a render conto ai cittadini di come spende le risorse. In particolare, a cadenza triennale, il Ministero dell'economia e delle finanze elaborerà un rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato illustrando la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni. Se sino ad oggi i Ministri delle finanze hanno proceduto a ridurre le spese o ad aumentare la pressione fiscale, oggi prevale l'idea che l'unico meccanismo per spendere meno è spendere meglio, ciò potrà avvenire con un miglioramento della legge di bilancio attraverso l'introduzione di un sistema di analisi e di valutazione delle *performance* unitamente all'analisi e alla valutazione della spesa cui è dedicato il Capo IV del provvedimento in questione. Per le ragioni sin qui illustrate, dichiaro quindi il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare. Signora Presidente, l'importante provvedimento che ci accingiamo ad approvare consentirà una gestione molto più semplice e trasparente dei conti pubblici. Evidenziamo in particolare tre aspetti positivi. Il primo è proprio la trasparenza: viene messo a regime il sistema approvato dal precedente Governo della suddivisione per missioni e programmi. Questo è molto importante perché si arriva ad una chiarezza delle scelte: rimane infatti lo stesso sistema di anno in anno e quindi è possibile valutare come il Parlamento va ad allocare le risorse,

avranno un chiaro obiettivo da portare a casa e sarà dunque più facile valutare l'operato sulla base degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Deve diventare sempre più un patrimonio comune il fatto che il problema vero è aggredire lo *stock* di spesa pubblica piuttosto che accapigliarsi sulla cosiddetta legge finanziaria. Anche se forse saremo noiosi, è bene

sono società perennemente in perdita che vivono del finanziamento da parte degli enti locali. È evidente a tutti che il confine con la pubblica amministrazione va considerato in una maniera piuttosto elastica o, meglio, nel caso di questi cosiddetti carrozzoni, è evidente che non sono mercato, ma Stato. Come risolvere il problema? Secondo noi è facile: basterebbe consolidare il bilancio delle aziende che non sono di fatto sul mercato. Facendo così, obbligheremmo gli enti locali a dismetterle immediatamente. Non si conclude tutto oggi in questa sede: questa legge avrà ulteriori affinamenti e modifiche nell'altro ramo del Parlamento.

è sicuramente un buono testo e un'ottima base di partenza con la giusta flessibilità per tenere conto anche delle altre importanti riforme che il Parlamento sta portando avanti. convintamente a favore di questa importante riforma.

perché la struttura del bilancio fissata da questa nuova legge di contabilità è quella articolata per missioni e programmi introdotta dal Governo Prodi e dal ministro Tommaso Padoa-Schioppa, che qui voglio ancora ringraziare per il lavoro svolto su questo punto in quella delicata fase. Il Governo in carica a questo proposito ha certamente un merito politico che voglio riconoscere apertamente, come spero venga riconosciuto - e lo è stato nella discussione che abbiamo svolto finora - il contributo determinante che l'opposizione

di buttare a mare il lavoro ingente che era stato svolto su questo tema nei dieci anni precedenti e che non aveva portato - questo era il limite politico gravissimo di quella lunga fase di discussione - all'approvazione di una nuova legge di contabilità. Se si arriva oggi ad un risultato positivo è perché non si è preteso di cambiare strada da parte dell'attuale maggioranza e dell'attuale Governo ricominciando tutto daccapo e perché l'opposizione non ha cambiato atteggiamento sulla base del fatto che nel frattempo da maggioranza è diventata opposizione sullo stesso argomento. Questo mi sembra il primo punto da sottolineare. In secondo luogo votiamo a favore perché gli strumenti fondamentali e i tempi della decisione di bilancio, così come sono definiti da questa nuova legge di contabilità, sono per l'essenziale quelli previsti dalla risoluzione approvata due anni e mezzo fa con i voti dell'allora maggioranza, cioè con i voti dei Gruppi del centrosinistra, a conclusione del confronto sviluppatosi per mesi - i colleghi Vegas e Azzollini lo ricorderanno - nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato nel corso di quella Una prima ragione del nostro voto favorevole è da rinvenirsi dunque nella linea di continuità che si può agevolmente tracciare tra questo disegno di legge, così come risulta alla fine delle votazioni in Commissione e in Aula, e le soluzioni di riforma della legge n. 468 del 1978 e delle parti relative dei Regolamenti parlamentari che il centrosinistra ha elaborato e proposto nel corso degli ultimi dieci anni. anni. Siamo un partito serio, voglio sottolinearlo ancora, e non modifichiamo le nostre idee sullo stesso tema a seconda della collocazione di minoranza o di Governo che ci capita di dover assumere. Una seconda ragione di favore è determinata dalla qualità e quantità degli emendamenti da noi presentati e approvati, prima in Commissione e poi ancora adesso, durante la lettura in Aula. L'intero titolo sulla trasparenza è stato da noi proposto e approvato,

E la conoscenza, signora Presidente, è il presupposto della decisione consapevole da che mondo è mondo. In secondo luogo, è frutto di un nostro emendamento l'introduzione della delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa che uniformerà, quando il decreto delegato sarà stato emanato, le nostre regole contabilistiche a quelle in vigore nei principali Paesi europei, cosicché aumenterà la possibilità di fare quella che gli economisti chiamano operazione di *benchmarking*, cioè l'operazione di comparazione alla dimensione, in particolare, dell'area dell'euro.

più responsabilità dei dirigenti pubblici nella gestione di ciascun programma di spesa. Il risultato complessivo sarà una migliore confrontabilità e una maggiore possibilità di introdurre indicatori di *performance* che consentano una lettura dell'efficacia e dell'efficienza della spesa, finalmente comparabile con quella di altri Paesi. In terzo luogo, è stato ancora un nostro emendamento a conferire maggiore profondità temporale alla Decisione quadro di finanza pubblica, il vecchio DPEF. Per un Paese che ha uno Stato indebitato come il nostro - anche se adesso siamo in buona compagnia su questo punto - si tratta di una acquisizione vitale:

l'ordine del giorno G100 pare molto ragionevole, al di là dell'aspetto tecnico del laboratorio che dovrebbe certificare.

13.100 è contrario perché mi sembra che la Commissione si sia concentrata molto sulle garanzie dei soggetti che hanno commesso i reati.

prevedeva la non utilizzazione e quindi la cancellazione dei profili del DNA soltanto a seguito di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. il disegno di legge e riprendendo anche elementi della discussione nel Senato, ha inserito tra le formule assolutorie che impongono la distruzione del campione anche «il fatto non costituisce reato» o «il fatto non è previsto dalla legge come reato». reato». L'emendamento 13.100 punta ad estendere la distruzione e comunque la non utilizzazione del campione a qualsiasi tipo di formula, anche di archiviazione e di proscioglimento, incluse quella di non imputabilità o di ritenuta non punibilità del soggetto accusato del reato. Questo crea un'anomalia nel sistema e, a nostro avviso, non va nella direzione del rafforzamento delle garanzie. Immaginiamo che ci sia un soggetto autore di un reato anche particolarmente grave, un omicidio o una violenza, che non abbia ancora compiuto l'età che permetta di essere anche solo parzialmente imputabile. L'impossibilità di utilizzare quel campione spingerebbe le forze di polizia comunque a cercare ipotetici autori del reato e a non avere un responsabile di fatto, anche se poi l'autore di fatto viene dichiarato esente da responsabilità perché non ha ancora compiuto gli anni. Questo crea uno squilibrio nel sistema e allo stesso modo in tutti i casi dai quali deriva la non imputabilità o non punibilità. A nostro avviso, quindi, la formulazione trovata dalla Camera è un corretto equilibrio tra le esigenze imprescindibili di garanzia e quelle di accertamento dei reati. Questo equilibrio verrebbe alterato dall'approvazione dell'emendamento 13.100, di cui comprendiamo l'intento garantista, ma forse rappresenta un eccesso di garanzie che va contro la

all'indicazione concernente l'articolo 425 del codice di procedura penale e al riferimento all'archiviazione del procedimento. In entrambi questi casi non si ha una chiusura definitiva del procedimento in quanto, sia in un caso, che nell'altro, con motivazioni e formalità diversificate, si potrebbe riprendere l'indagine e quindi potrebbe essere necessario utilizzare i dati del DNA individuati e raccolti a suo tempo. Per questa parte quindi sicuramente non possiamo essere d'accordo, anche se per il resto l'emendamento poteva essere convincente. Per queste ragioni ci asterremo, anche perché come Partito Democratico riteniamo fondamentale che il Trattato di Prum, che trae origine, all'epoca, dai lavori del ministro dell'interno Amato e da un insieme di articoli

Alla casistica indicata dal signor Sottosegretario si aggiunga il caso di un indagato

il profilo ricavato dal campione biologico potrebbe dare una conclusione alla vicenda. Riteniamo che le integrazioni al provvedimento, apportate dalla Camera con l'inserimento di altre due formule assolutorie, abbiano dato ampia garanzia

Il prossimo ed ultimo tassello di questo pacchetto lo affronteremo la prossima settimana. Otto provvedimenti in poco più di un anno dimostrano nei fatti che questo Governo e il ministro Maroni si siano dati particolarmente da fare su questo obiettivo della sicurezza.

il lavoro parlamentare e il modo di scrivere le norme che hanno a che fare con la sicurezza dei cittadini e, al tempo stesso, con le garanzie per i cittadini. Sono entrambe annotazioni positive relative a questo provvedimento. La prima ha a che fare con la circostanza che su questo provvedimento, che peraltro viene da lontano viene dal lavoro del ministro Amato e da progetti di legge di diverse forze politiche che hanno trovato una convergenza significativa nel testo finale,

i diversi punti di vista e senza dimenticare le diverse prospettive su questi temi, ma al tempo stesso tenendo presente il fatto che su certi argomenti, come questo, è importante - se non fondamentale - che vi sia una significativa convergenza e un lavoro parlamentare civile,

Questo sul metodo. ulteriori affinamenti - sia un buon provvedimento. In questo caso ci troviamo di fronte ad un sano equilibrio tra garanzie per i cittadini e tutela della collettività. Non credo - davvero non c'è nessun tono polemico in quello che sto per dire

sia soddisfatta unitamente a quella della sicurezza dei cittadini. Detto ciò e ritenendo del tutto superfluo entrare nel dettaglio di alcune singole disposizioni, ribadisco che il Partito Democratico voterà a favore.

la maggioranza e il Popolo della Libertà dimostrano con quale efficienza e capacità portano all'approvazione il Trattato di Prum, sottoscritto il 27 maggio 2005. Sono state individuate soluzioni molto importanti per il prelievo dei campioni biologici, superando alcune criticità sollevate da alcune sentenze della Corte costituzionale e credo che si sia raggiunto un ottimo equilibrio, in considerazione dei diritti di *habeas corpus* ma anche della tutela dei diritti connessi con l'articolo 32 della Costituzione. Pertanto, i prelievi coattivi godono nel nostro Paese di garanzie molto significative finalmente, con l'istituzione della banca data del DNA, le Forze di polizia del nostro Paese possono cooperare e rafforzare il secondo pilastro delle politiche europee e del Trattato di Schengen, perché sarà possibile scambiare i dati relativi ai profili biologici Grazie a tutti. in materia di terrorismo internazionale e di gravissimi reati, ma anche in materia di ordine pubblico e di grandi manifestazioni internazionali. Tale provvedimento corrobora le altre leggi approvate lo scorso anno, in particolare il decreto-legge sulla sicurezza. La prossima settimana approveremo l'atto Senato n. 733 in materia di sicurezza dei cittadini, portando a compimento, dopo solo un anno dall'avvio della XVI legislatura, il programma delineato in campagna elettorale, ossia il rafforzamento dei livelli di sicurezza dei cittadini.

pertanto che il nostro Paese dimostri anche a livello internazionale quale sia l'efficienza del Gabinetto Berlusconi e della XVI legislatura. Concludo con due ulteriori riflessioni sul fatto che il disegno dà la possibilità di approvare a brevissimo giro anche la legge sulle persone scomparse, e per la prima volta viene istituito il ruolo tecnico della Polizia penitenziaria, una rivendicazione dal Corpo lungamente richiesta. La conclusione non può che essere che il Gruppo del Partito della Libertà vota convintamente tale provvedimento, perché anche da questo punto di vista i risultati del contrasto e della lotta alla criminalità ci danno già ragione: c'è già un abbattimento del numero dei reati denunciati quest'anno. Dalla politica delle parole noi siamo passati alla politica dei fatti.

(che poi è stata interrotta) e che la Camera aveva approvato. Ora noi sottolineiamo la necessità per il Parlamento italiano di provvedere alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Ricordo che il testo all'esame dell'Assemblea è stato approvato all'unanimità; dopodiché vi è stato un testo unificato elaborato da un apposito Comitato ristretto infine, alla conclusione dei lavori delle Commissioni, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1594, che dispone l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione recando norme di adattamento

come è noto a tutti, il 9 dicembre del 2003, oltre cinque anni fa, a Merida, lo Stato italiano ha sottoscritto la Convenzione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite

Il Comitato costituito *ad hoc* fu deputato alla redazione del testo e alla sua negoziazione fino all'approvazione che avvenne nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a Vienna nell'ottobre del 2003.

tra l'altro come seguito della Convenzione di Palermo sul crimine transnazionale, dunque dopo avere partecipato ai lavori di Palermo. In quella sede si ritenne insufficiente la previsione in materia penale ed in materia di prevenzione nella lotta contro la corruzione, poiché la corruzione dei pubblici ufficiali veniva esaminata soltanto per aspetti collegati al crimine trasnazionale; quindi era una prospettiva assolutamente riduttiva.

che copre alcuni punti fondamentali della lotta alla corruzione e per la verità - mi permetto di dire, signora Presidente - non mi meraviglia che non interessi, visto quello che sta accadendo in questo momento storico in materia di legislazione.

a rafforzare la cooperazione internazionale e la lotta contro il riciclaggio. Costituisce quindi per noi un'ottima base per continuare quel lavoro che alla delegazione italiana veniva riconosciuto come un importante contributo prestato dal nostro Paese, che si era specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione, in particolare nel periodo di contrasto a Tangentopoli. La firma di questa Convenzione dovrebbe comportare quindi contemporaneamente alcune garanzie, che ritengo indispensabili nel momento in cui vogliamo ratificare una Convenzione di questo rilievo. riferisco all'indipendenza dell'organo deputato ad assicurare il rispetto delle previsioni: ho ritenuto di non presentare un emendamento in materia, proprio per evitare che si fermasse l'*iter* dell'approvazione, ma non vi è dubbio che nel momento in cui dovessero essere reperite le risorse finanziarie - perché di questo stiamo parlando - lo Stato italiano dovrebbe assicurare la presenza di un organo indipendente.

*(PD)*. Sorprende che in questo momento in cui stiamo per ratificare uno strumento così importante vi sia un indebolimento degli organi e degli strumenti legislativi e del conseguente contrasto giudiziario alla corruzione. In particolare, mi riferisco al disegno di legge governativo sul nuovo processo penale

ancorare questi strumenti a determinati presupposti giuridici, alterando le regole del sistema e togliendoli ad un pubblico ministero specializzato (che dirigendo effettivamente la polizia giudiziaria deve utilizzare in questo campo tutti gli strumenti più adeguati,

questo, infatti, rappresenta uno sviluppo logico rispetto alla Convenzione sulla corruzione: non voglio richiamare la relazione introduttiva, che tra l'altro i colleghi relatori hanno svolto benissimo, ma anche lo stesso Governo, nel presentare il disegno di legge che poi è stato unificato, sostanzialmente richiama normative e direttive europee e internazionali che sono alla base delle nuove norme sull'autoriciclaggio.

e per la rapidità con cui maggioranza e opposizione hanno raggiunto al loro interno un accordo, nella comune consapevolezza che il tempo dei rinvii era ormai esaurito. Sono trascorsi ormai sei anni dall'adozione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della presente Convenzione e quasi quattro anni dalla sua entrata in vigore. Non era dunque accettabile che il Parlamento italiano continuasse a sottrarsi a questo dovere: il dovere di contribuire in maniera più incisiva alla lotta alla corruzione, almeno sul piano internazionale. alle considerazioni, nel nostro Paese stiamo arrivando a una resa incondizionata in termini di corruzione.

la Corte dei conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha evidenziato un quadro di corruzione ampiamente diffusa nel nostro Paese, con profili di patologia allarmanti nel settore dei lavori pubblici, delle pubbliche forniture e in materia sanitaria. In particolare, risultano in aumento le condanne per danni materiali e per danni all'immagine della pubblica amministrazione pronunciate dalla Corte dei conti in seguito al pagamento di tangenti durante la stipula dei contratti. Sempre la Corte dei conti, infine, ha rilevato un sistema di controlli insufficiente, scarsamente efficace e foriero di ben pochi effetti concreti (è questa una valutazione su cui tornerò tra qualche momento). Anche la cronaca politica locale ha registrato, da settembre a oggi, gravi e numerosi episodi o fondati sospetti, di corruzione all'interno della pubblica amministrazione. Per dare esecuzione e ratifica alla Convenzione dell'ONU, il testo unificato uscito dal lavoro delle Commissioni prevede all'articolo 6

Per amore di verità e chiarezza, vorrei qui ricordare i limiti e i risultati raggiunti dall'estate scorsa dal nuovo ufficio, battezzato SAeT creato nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica lo scorso ottobre dopo la soppressione dell'Alto commissario e in seguito a una conferenza stampa congiunta tra il Presidente del Consiglio dei ministri e Brunetta. Onorevoli colleghi, si tratta di un organo che conta meno di 20 dipendenti (laddove a Singapore sono oltre 800) e che ha a disposizione una sola autovettura con oltre 100.000 chilometri e mezzi assai inadeguati a svolgere il compito di contrasto alla corruzione e agli illeciti della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale. In quasi un anno di vita questo nuovo ufficio ha stipulato all'incirca una dozzina di protocolli e partecipato ad alcuni incontri internazionali. Non un'azione concreta, non un'indagine fruttuosa: un fallimento non imputabile al personale in servizio, che in larga parte è lo stesso che ha efficacemente supportato l'attività dell'Alto commissario, che fu abolito, tra l'altro, per risparmiare 5 milioni l'anno (menzogna, questa, perché già il precedente Governo ne aveva ridotto il *budget* a un milione di euro). Sicuramente i viaggi all'estero dei vertici dell'ufficio e gli stipendi dei dipendenti sono stati pagati, mentre nessuna risorsa è stata concessa alla finalità prioritaria del nuovo ufficio, ossia l'operatività sul fronte della corruzione.

In esso si stima che la corruzione nel sommerso sia pari almeno a 50-60 miliardi di euro l'anno. Una cifra che, se attendibile, significa una tassa-corruzione pari a 1.000 euro a testa, compresi i neonati, oltre il danno sul piano morale e della fiducia. Gli elementi necessari indicati dal SAeT per una vera azione sono la volontà politica, la pressione dell'opinione pubblica, nuovi strumenti per analizzare e trattare il rischio, strumenti al momento inesistenti. Né d'altro canto si può rinunciare alla prevenzione ed affidarsi al lavoro delle forze dell'ordine. Queste infatti - è bene ricordarlo - già faticano a smaltire il lavoro quotidiano e difficilmente possono dedicarsi alle complesse indagini investigative che richiede una seria azione di contrasto alla corruzione. A onor del vero, onorevoli colleghi, occorre ricordare che anche l'alto commissario, organo facente capo alla Presidenza del Consiglio, soffriva di una grave carenza di mezzi, pur senza raggiungere questi straordinari eccessi. La pianta organica allora prevedeva oltre 80 persone: una squadra esigua rispetto all'entità della missione, ma sufficiente a mettere a segno qualche risultato concreto. Per limitarci all'anno e mezzo precedente la sua soppressione, voglio qui ricordare l'indagine sulla sanità in Calabria; l'indagine che ha messo in evidenza le gravi carenze dell'ospedale Umberto I di Roma; l'indagine relativa alla ASL Napoli 5, che ha fatto emergere profili di possibile infiltrazione della criminalità organizzata; l'attivazione di un numero verde che, consentendo ai cittadini la denuncia degli illeciti dietro garanzia di anonimato, è divenuto significativo punto di riferimento per l'intera comunità su questo delicato terreno e che ovviamente è stato disabilitato dal nuovo ufficio. Oltre naturalmente alla sigla di numerosi protocolli d'intesa con enti pubblici, dal Ministero per le riforme a quello delle infrastrutture, dalla Corte dei conti all'Agenzia delle entrate. La decisione del Governo di restringere ulteriormente il campo d'azione dell'ufficio preposto al contrasto della corruzione, onorevoli colleghi, ha inferto un grave colpo al Paese essendo questo male, quello della corruzione, che Transparency International definisce abuso di pubblici uffici per il guadagno privato. Pratica altamente nociva sotto tutti i profili, pratica dunque che mina la democrazia alle sue fondamenta, come sottolineato dalla collega Biondelli in una interrogazione cui ovviamente mai è stata data risposta. L'auspicio è quello e lo esprimo in questa sede in questo momento - che venga data esecuzione ad una Convenzione delle Nazioni Unite sul tema e che la volontà politica inverta la propria rotta ed inizi a considerare il contrasto alla corruzione a tutti i livelli una battaglia civile irrinunciabile, che non può combattersi solo a parole.

Lo strumento che ci accingiamo ad approvare promuove e rafforza il contrasto alla corruzione o ai fenomeni ascrivibili al mondo della corruzione. Incentiva la cooperazione internazionale nella lotta a questi fenomeni, valorizza la trasparenza, la correttezza, l'integrità e la buona fede nella gestione degli affari. Abbiamo ormai un'economia

individuarsi aree di nuova e pesante corruzione, e ce ne è tanta.

anche aiutati nell'individuazione di filoni di contributi per diverse decine di miliardi di euro da uffici della Comunità europea. È un grosso problema. Voglio rammentare uno degli ultimi casi all'esame della magistratura: la realizzazione in Calabria del complesso "Europaradiso", un intervento da 7 miliardi di euro, che prevedeva un intervento violento sul territorio (40.000 posti letto) in una zona protetta, e che è stato reso possibile solo perché - così recita l'accusa - un funzionario della Comunità europea aveva fatto sparire la documentazione riguardante la sottoposizione dell'area individuata al vincolo di protezione ambientale. quindi il problema ed allora lo strumento era necessario, perché ormai la corruzione nasce anche fuori dai nostri confini. di un intervento assolutamente necessario, nella speranza di avere nel nostro Paese un'economia pulita.

dell'agente attivo corruttore, che approfitta del proprio *status* per imporre il pagamento di un prezzo non dovuto. dovuto. Sappiamo che a livello europeo si tenta o si è optato per comunque rientrare la concussione nell'alveo della corruzione, ma il nostro sistema oggi prevede

soltanto ad una delle due ipotesi di reato previste dal nostro sistema. Di fronte a questa incomprensibile scelta del Governo noi andremo sicuramente

di ratifica e quindi di modifica del codice penale nella sua completezza, ma così come oggi è il codice penale. Attendiamo pertanto con curiosità di sapere dal Governo quali sono le ragioni per cui intende far sparire la concussione, reato oggi esistente, e privare questa tipologia di grave condotta delittuosa della copertura di sanzione

a ratificare dandole esecuzione e quindi introducendola nel nostro ordinamento per la sua applicazione. Ricordava infatti la collega che tale Convenzione è stata adottata nel lontano 31 ottobre 2003 dall'Assemblea generale dell'ONU

quindi un processo dovuto - ben si ricordava l'interruzione della precedente legislatura - che si compie soltanto oggi, cioè nel 2009, a quasi sei anni di distanza dall'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite.

in questo caso della comunità internazionale. Il provvedimento consta sostanzialmente di due parti. La prima integra

si autorizza la ratifica e si dà l'ordine di esecuzione. Dall'articolo 3 in avanti si introducono norme di recepimento, di modifica e di adeguamento interno rispetto alla normativa del codice penale in particolare, e del codice di procedura penale.

All'articolo 3 si fa riferimento alla disciplina relativa alla prevenzione, alle indagini e ai procedimenti riguardanti la corruzione, i sequestri, la confisca e la restituzione dei proventi dei reati ad essi connessi.

nella direzione della prevenzione della corruzione, della repressione delle condotte criminose e della cooperazione internazionale in materia, che credo siano parte importante dell'atto

di confisca adottati all'estero. È una fattispecie complessa, che però consente allo Stato straniero che ha posto in essere un provvedimento di natura

nel provvedimento con il quale delibera il riconoscimento della sentenza o del provvedimento di confisca, a ordinare contestualmente la devoluzione delle cose confiscate. Si è detto che si tratta di un ragionamento tecnico

descrizione generale, di un invito alla cooperazione internazionale, ma poi la cooperazione si misura nell'efficacia e nell'introduzione di norme tecniche che consentano quei procedimenti. Nell'articolo 6 - lo ricordavo già prima - è prevista l'istituzione dell'Alto Commissario, che il Governo nel suo disegno di legge

che con i suoi contenuti tecnici fissa un punto più avanzato nella lotta alla corruzione dentro la cooperazione internazionale, rappresenta *(PdL)*. Signora Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto hanno sottolineato come i tempi del nostro lavoro legislativo siano talvolta tremendamente in ritardo. l'occasione delle ratifiche dei trattati internazionali è quella che maggiormente induce questo tipo di considerazione. Qui è stato ricordato che siamo a sei anni dalla Convenzione e a quattro anni

D'altro canto, però, non mi è sfuggito, avendo ascoltato gli interventi dei colleghi, come da parte di senatori dell'opposizione si chiedano Grazie a tutti.

sulla corruzione è generico e si presta ad alcuni argomenti e sentimenti fuori tempo e fuori tema, come mi sono sembrati quelli della collega Della Monica.

considerata anche in relazione a un'ottica di mantenimento delle relazioni internazionali con i Paesi membri delle Nazioni Unite.

se vogliamo la società aperta - è una formula liberale di Popper che forse risale ad Hayek e Mises

si può anche fare - mi pare l'abbia fatto la senatrice Della Monica - qualche riferimento alle cronache nostrane di Tangentopoli. Attenzione però a non guardare soltanto

di tipo sovranazionale, che si inserisce nel mondo della *civil society*, della società aperta e delle sue regole negli affari internazionali.

giudizi su provvedimenti legislativi quali la riforma del processo penale o il provvedimento in materia di intercettazioni, che credo sia già all'attenzione dei colleghi della Commissione giustizia e bussa, se non per la prossima settimana, per quelle successive, alle porte dell'Aula. Credo che dobbiamo mantenere la discussione su un profilo più alto, come ci invitava a fare l'ultimo intervento con una puntuale ricostruzione degli articoli del disegno di legge. legge. A proposito di questi articoli, vorrei riprendere, proprio per attenuare, se ci riesco, le perplessità, a mio giudizio un po' fuori tema e un po' fuori tempo, della senatrice Della Monica, come quell'articolo 6,

meno pessimismo di quello con il quale il senatore Serra ne ricostruiva precedenti e predecessori. rispetto ad impropri richiami a cronache e commenti tangentopolitani, voglio ricordare che all'articolo 6, secondo comma, si dice che a questo organo vogliamo assicurare autonomia ed indipendenza nell'esplicazione dell'attività. Sono termini che la nostra Costituzione adopera Grazie a tutti. è stata interpretata nel modo meno liberale e più corporativo, laddove il dettato della nostra Costituzione era all'autonomia e all'indipendenza

all'autorità nazionale che andremo a costituire in base all'articolo 6 di onorare lo spirito che portò nel 2003 a quella Convenzione internazionale. La ringrazio del richiamo che mi fa alla conclusione. La mia conclusione è perfettamente in linea con il punto di partenza: condivido anch'io, con il relatore, la necessità di un'adesione rapida e di un'approvazione da parte di quest'Aula. E se ho voluto rispondere ad alcune sollecitazioni del dibattito è proprio per ritornare all'essenzialità

in modo che il privato che corrompe i pubblici ufficiali stranieri o appartenenti a organizzazioni internazionali non possa invocare l'induzione esercitata dal pubblico ufficiale al fine di vedere esclusa la propria responsabilità. Il Governo, dopo aver ascoltato alcune valutazioni, ritiene di dover

*(PdL)*. Signora Presidente, tenuto conto che giovedì scorso si è svolto un incontro tra il Governo, la FIAT e i sindacati sulla questione della chiusura o del mantenimento in vita degli stabilimenti in Italia,

deportazione di cani che sta per avvenire in Basilicata. Prima il rischio era che andassero in Campania, in un canile che è stato chiuso

finestra"), presentata il 20 maggio scorso, invece della risposta del Ministro dell'economia, ho ricevuto una risposta dalla Banca d'Italia tramite un quotidiano economico che probabilmente considera un suo

signora Presidente, colleghi, comprendo l'imbarazzo della Banca d'Italia e del suo direttore generale Fabrizio Saccomanni, che aveva dato autorizzazione al gruppo Delta nonostante il parere di un autorevole giurista inviato nel 2007, prima dell'autorizzazione alla Banca d'Italia, che denunciava un controllo occulto di Delta e Cassa di Risparmio di San Marino. Ma se facciamo passare che le risposte alle interrogazioni parlamentari invece che dai Ministri competenti vengano date sui giornali, il cui servilismo ai potentati economici peraltro è acclarato, sviliamo la nostra funzione e la stessa dignità del Parlamento e dei parlamentari. Intervengo, quindi, affinché la Presidenza stigmatizzi questi comportamenti e queste

Signora Presidente, anch'io desidero sollecitare, con ampio ritardo rispetto ad altri miei colleghi, una mia interrogazione indirizzata al ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali finestra"), in merito ad un eventuale conflitto di interessi che potrebbe sorgere visto il legame di parentela che lega il titolare del Dicastero e il direttore generale di Farmindustria, dottoressa Enrica Giorgetti. Da un anno, precisamente dal 1° luglio 2008, è stata presentata questa interrogazione al Ministro, anche in forma scritta

prego la Presidenza di questo Senato di tutelare la dignità dei parlamentari e di un senatore che ha tutto il diritto di avere una risposta da parte del Ministro. *(Applausi del